di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo

nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

il provvedimento fu riproposto quindi nella XV legislatura, nel corso della quale furono presentati disegni di legge tanto alla Camera quanto al Senato. L'*iter* legislativo in materia iniziò alla Camera dei deputati e fu approvato un testo che demandava a un decreto del MIUR la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi e delle modalità di espletamento di corsi di formazione e tirocinio ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia da parte dei laureati in scienze motorie. Quando il testo pervenne all'esame del Senato, quest'ultimo ebbe la tentazione di approvare un emendamento con il quale si abrogava in maniera secca l'equipollenza delle due lauree ma, in un'ottica di mediazione con l'altro ramo del Parlamento, fu convenuto di mantenere aperta la possibilità di conseguire il diverso diploma di laurea nel rispetto della normativa vigente. Più precisamente, il Senato voleva che i laureati in scienze motorie fossero sottoposti a una selezione per l'accesso a fisioterapia, naturalmente nell'ambito del fabbisogno In effetti, l'equipollenza disgiunta dalla selezione avrebbe significato un modo surrettizio per aggirare la programmazione degli accessi previsti dalla legge. La Camera rifiutò tale modifica e pertanto il problema si ripropone

l'accesso al corso di fisioterapia nel limite dei posti programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione; la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente. A dire il vero, in Commissione è stata forte la tentazione di modificare ancora il testo nel senso di approvarlo nella sua forma originaria, quella che prevede l'abrogazione secca. Poi, in seguito a un'audizione in 7a Commissione con il ministro Fazio, e riflettendo sul fatto che modificandolo ulteriormente probabilmente questo testo non avrebbe avuto più conclusione perché sarebbe stato fermato nell'altro ramo del Parlamento, abbiamo ritenuto essere prevalente

che dispose l'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Anche in Commissione sanità del Senato, in particolare, la preoccupazione espressa era riferita all'esigenza primaria

Riteniamo però che i diritti di queste categorie debbano essere salvaguardati, sempre nel quadro delle tutela delle persone più deboli. La soluzione che oggi emerge tenta di coniugare questi due aspetti, anche perché eliminare l'equipollenza corrisponde all'esigenza vera di non sovrapporre percorsi di laurea molto diversi. Nello stesso tempo, attraverso una delega all'Esecutivo, si rinvia ad un atto congiunto del Ministro dell'istruzione e dell'università di concerto con il Ministro della salute adottare un decreto che renda possibile il conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e per gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie.

che le preoccupazioni che già abbiamo manifestato nei dibattiti precedenti, sia in quella stessa Commissione che nelle altre, trovino appropriato

Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, sono quasi incredulo che la vicenda relativa all'equipollenza del diploma di laurea in fisioterapia a quello in scienze motorie sia ad un passo dall'epilogo.

a trovare una soluzione ad un'ingiustizia perpetrata ai danni dei laureati in fisioterapia, prima, ai danni degli stessi laureati in scienze motorie, dopo, e ai danni, infine, ma non certo in ordine di importanza, della collettività tutta. Lo premetto, colleghi, se non altro perché, almeno per la mia coscienza, vorrei continuare ad essere chiaro ed onesto su questo annoso problema. La soluzione propostaci dai colleghi della Camera dei deputati non è, né ad opinione mia, né del mio Gruppo, ottimale: un legislatore attento avrebbe potuto fare prima e meglio. In ogni caso, prima di passare in rassegna le motivazioni sottese a questo nostro intendimento, voglio altrettanto chiaramente affermare che sia io che il mio Gruppo voteremo a favore del provvedimento in questione nel testo in cui ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Voteremo a favore perché vogliamo fermamente che questa diventi presto la legge per ridare giustizia e dignità al meritorio impegno di decine di migliaia di laureati in fisioterapia. Questo potrà accadere a breve grazie ai colleghi che contribuiranno a formare una maggioranza su questo testo, qualunque sia lo schieramento di appartenenza. un atto di giustizia nei confronti dei laureati in fisioterapia senza, al contempo, prevedere alcuna prevaricazione dei diritti già riconosciuti nel contesto normativo ai laureati in scienze motorie, veri grandi sconfitti, non dalla legge che si sta per approvare, ma dalla presa in giro che il famigerato articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 250 del 2005 ha perpetrato ai loro danni per ben cinque anni. Ma se, come si dice, il tempo è galantuomo, come dovrebbe essere in questo caso - lo vedremo fra poco - spero fortemente che anche per loro, per le altrettante decine di migliaia di studenti che si sono laureati e si stanno laureando in scienze motorie, si troverà - ne sono convinto - una soluzione, uno sbocco occupazionale certo e garantito. Voglio a questo punto, colleghi, soffermarmi solo per qualche minuto sulla genesi di questo provvedimento. Con un *blitz*, con una porcata, un atto, comunque lo si voglia definire, inqualificabile lo dico solo per dovere di cronaca e non per attaccare i colleghi di una parte o dell'altra - negli ultimi giorni di legislatura - era il febbraio del 2006 - si pensò bene di presentare un emendamento ad un decreto-legge (il decreto-legge n. 250 del 2005) allora con il quale veniva introdotto, nella disattenzione più generale, l'ormai tristemente noto articolo 1-*septies*. A riprova di quanto detto, la maggioranza di allora, accortasi del fattaccio come ha detto il collega Bevilacqua - approvò un ordine del giorno con il quale impegnava il Governo a cancellare questo obbrobrio legislativo. Pochi mesi dopo, con le Camere ed il Governo nuovo, è iniziata una lunga battaglia di posizionamento dei partiti, dei Gruppi parlamentari, dei singoli parlamentari all'interno dei Gruppi. Una battaglia nascosta, sotto traccia, su una questione che non sarebbe mai, e ripeto mai, dovuta durare tutto questo tempo. Colleghi, più del fatto che sia stata apportata, con una furbata, una modifica impropria all'ordinamento giuridico, dopo cinque anni dall'accaduto (che corrispondono peraltro ai miei cinque anni di attività parlamentare) la cosa che più mi ha fatto riflettere e mi ha fatto dispiacere è stato proprio questo comportamento ondivago, ambiguo, non corretto né di fronte agli elettori né di fronte ai laureati di entrambe le categorie. Comportamento ondivago, sia chiaro, registrato in entrambi gli schieramenti, in entrambe le legislature. Spero che sia arrivata l'ora della soluzione. Una soluzione che, come ho già detto, non è la mia preferita, ma è pur sempre una soluzione. E, invece di convincermi della necessità di continuare a combattere con il coltello tra i denti a difendere una enunciazione di principio secca, sono disposto a fare anche un piccolo passo indietro, accettando la formulazione approvata dai colleghi della Camera, purché questa situazione di *impasse* trovi fine. Senza tediare i colleghi tutti con l'elenco degli atti ed i passaggi amministrativi e giudiziari che questa ignobile "normetta" ha causato in questi anni, vorrei solo accennare alle motivazioni che mi hanno portato, insieme al Gruppo dell'Italia dei a sposare questa battaglia, anche e soprattutto per dovere di chiarezza nei confronti dei laureati in scienze motorie. Mi rivolgo ai colleghi che non provengono da questo settore, mi rivolgo ai tanti colleghi in quest'Aula che esercitano la professione medica e quella di docenti all'università. Il corso di laurea in fisioterapia è uno dei corsi di laurea attivati, su tutto il territorio nazionale, là dove ci sono delle facoltà di medicina che, garantendo l'espletamento dei test per il numero chiuso, formano gli studenti, in numero programmato appunto, su una professione sanitaria, qual è la fisioterapia. Senza nessun intento polemico nei confronti di chi tenta di difendere posizioni indifendibili, le professioni sanitarie sono tutte quelle figure necessarie e presenti per il normale svolgimento del Servizio sanitario nazionale.

indifendibili, le professioni sanitarie sono tutte quelle figure necessarie e presenti per il normale svolgimento del Servizio sanitario nazionale. Tra queste, nel novero delle professioni riabilitative, c'è, appunto, la fisioterapia. Scienze motorie è invece la denominazione di un corso di laurea o di facoltà universitaria. Tale denominazione è nata in sostituzione del vecchio ISEF (Istituto superiore di educazione fisica statale), a seguito del decreto legislativo dell'8 maggio 1998, n. 178. In base al suddetto decreto, all'articolo 2, comma 7, si legge testualmente: «Il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio di attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia, e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni». E sin qui è tutto chiaro, e soprattutto è corretto l'operato del legislatore di allora. pur conscio che alcune materie oggetto dello studio di questi ragazzi potessero sembrare, ed in alcuni casi essere, uguali a quelle degli studenti dei corsi abilitanti alle professioni sanitarie - ha correttamente distinto la formazione di questi studenti da quella dei fisioterapisti, i quali - voglio ribadirlo - sono professionisti che curano la patologia, la malattia: non curano cioè il benessere della persona, come in qualunque centro massaggi, ma curano il malessere. di laurea in scienze motorie è» (magicamente diventato) «equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituire con decreto ministeriale, presso le università». A seguito dell'incapacità della maggioranza di centrosinistra di cancellare questa norma vergognosa, dopo mille passaggi parlamentari su «abrogazione secca sì, abrogazione secca no», «comma aggiuntivo o non comma aggiuntivo», dopo alcune pronunce dei tribunali, è arrivato un decreto ministeriale del 24 febbraio febbraio 2009 per disciplinare il modo in cui questa equipollenza doveva avvenire. Fortunatamente, l'imbarazzo del Ministero della salute circa questo decantato fabbisogno in soprannumero di laureati in scienze motorie ha evitato danni peggiori. Venendo a questa legislatura, colleghi, sin da subito mi sono impegnato per percorrere la scelta iniziale dell'abrogazione secca del provvedimento, ma, come sapete, alla Camera anche questa volta hanno rioptato per una formulazione ampia, con due commi aggiuntivi, che prevedono un decreto che tracci nuovamente le linee per il riconoscimento dei crediti formativi per gli studenti ed i laureati in scienze motorie - ovviamente ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia - che dovranno comunque superare le prove selettive previste per accedere ai posti programmati dal Ministero della salute. salute. Colleghi, questo compromesso era stato già approvato all'unanimità in questo ramo del Parlamento anche nella scorsa legislatura. Come correttamente affermato in varie occasioni dal relatore, collega Bevilacqua, nella scorsa legislatura - e se mi permettete anche in questa - il nodo vero stava nella scelta del Senato di sottoporre i laureati in scienze motorie ad una selezione per l'accesso a fisioterapia nell'ambito del fabbisogno programmato, in conformità all'ordinamento vigente. L'Italia dei Valori ha sempre reputato, infatti, che l'equipollenza disgiunta dalla selezione avrebbe rappresentato un modo surrettizio per aggirare la programmazione prevista dalla legge proprio per questo diploma di laurea. La Camera allora rifiutò questa proposta e non approvò la legge, ma questa volta fortunatamente ha compreso le nostre ragioni e speriamo di chiudere qui la vicenda. Oggi tocca a noi chiudere una volta per tutte questo contenzioso. La 7a Commissione, presieduta dal collega Possa, ha approvato all'unanimità, in prima lettura, il disegno di legge di cui sono primo firmatario e, quasi all'unanimità anche in questo secondo passaggio, sul testo modificato dalla Camera ha dato mandato al relatore di riferire all'Aula.

perdonatemi, colleghi - che ratificare quanto ci arriva dai colleghi di Montecitorio, perché è ora che i laureati in queste due professioni possano ritrovare la serenità e la certezza di un percorso formativo, prima, e poi professionale certo e non truffaldino, come quello che si è voluto far intravedere ai pur meritevolissimi laureati in scienze motorie. Sia chiaro, Presidente - e con questo concludo - che l'Italia dei Valori non è contro gli studenti e i laureati in scienze motorie. Non lo siamo mai stati e non lo saremo mai: abbiamo solo lottato, come chiunque altro avrebbe dovuto fare, per evitare che con una legge si potesse di fatto agevolare l'esercizio abusivo della professione sanitaria. Per quanto riguarda poi il percorso formativo e gli sbocchi professionali dei laureati in scienze motorie, con lo stesso spirito battagliero e con la voglia di trovare una soluzione formativa, e soprattutto lavorativa, a decine di migliaia di laureati ex decine di migliaia - ho presentato un disegno di legge (Atto Senato n. 796) contemporaneamente al disegno di legge in questione, misteriosamente fermo, però, in Commissione. Il disegno di legge in questione è diretto a fornire competenze professionali relative alla progettazione ed alla gestione di attività motorie di carattere educativo, ludico o sportivo, finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e al recupero delle capacità motorie e del benessere psicofisico ad esse correlato, obbligando le strutture che ospitano dette attività a dotarsi della direzione responsabile di un laureato in scienze motorie. Io invito i colleghi ad andare a recuperare il testo di questo disegno di legge e vorrei che qualcuno, anche nel caso non lo abbia condiviso appieno, mi spiegasse perché esso, dopo essere stato calendarizzato per ben quattro volte in Commissione in poco più di un mese nel 2008, si è letteralmente insabbiato. Ad ogni modo, colleghi, questo non è il momento delle recriminazioni o di intestarsi i meriti politici di un traguardo ancora da raggiungere. Non abbiamo in questa fase bisogno di medagliette. Questo è il momento di ristabilire la legalità all'interno del contesto normativo nazionale di settore. Poi, molto presto per quanto mi riguarda, come ho detto all'inizio di questo mio intervento, il tempo sarà galantuomo anche nei confronti dei laureati in scienze motorie, e io rappresento qui, ora, tutta la disponibilità del Gruppo dell'Italia dei Valori a costruire insieme la soluzione lavorativa anche per questi meritevoli studenti e per i già laureati. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci accingiamo a discutere in quest'Aula del Parlamento ha vissuto un travaglio lunghissimo, iniziato nella XIV Legislatura. L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha previsto l'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia, previa definizione di un decreto ministeriale per dettarne le modalità applicative. Nel corso dell'esame in seconda lettura, la Camera dei deputati si è resa conto dell'inopportunità di questa disposizione, che oltre ad apparire contraria alla Costituzione, alle direttive europee e a ogni altra normativa vigente in Italia, era in stridente contrasto con il testo della legge 10 febbraio 2006, 2006, n. 43, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali, approvata definitivamente il 24 gennaio 2006, pochissimi giorni prima della legge di conversione del citato decreto-legge n. 250 del 2005, dalla stessa Camera dei deputati. Più specificamente, il citato articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 250 del 2005 presenta evidenti profili di incostituzionalità in quanto interviene con una norma di dettaglio sull'esercizio delle professioni sanitarie, materia in cui, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, allo Stato è demandata la determinazione dei principi, mentre spetta alle Regioni la potestà legislativa di dettaglio. La competenza regionale è stata confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 424 del 2005 e appare rispettata nell'assetto normativo delineato dalla citata legge n. 43 del 2006, sulle professioni sanitarie, che prevede accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le norme dell'articolo 1-*septies* presentano poi evidenti profili di contrasto con le disposizioni dell'Unione europea sulla formazione universitaria e con la recente direttiva europea 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e forti contrasti con il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, articolo 2, comma 7, che disciplina il profilo dei laureati in scienze motorie, non abilitandoli all'esercizio di attività sanitarie. Il corso di laurea in scienze motorie, d'altronde, non è sicuramente aderente al profilo professionale approvato dal decreto del Ministro della salute per la formazione dei fisioterapisti. Il predetto articolo di legge, qualora non fosse abrogato, renderebbe inefficace la programmazione annuale nazionale per l'accesso ai corsi di laurea in fisioterapia, disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base di dati regionali. Infine, in via generale, si finirebbe di fatto per affidare la salute dei cittadini a personale non sanitario. Con il nuovo testo, si abroga l'equipollenza della laurea in scienze motorie con il diploma di laurea in fisioterapia, attribuendo al Ministro competente il compito di definire la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi; l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione; la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente. Durante la discussione in 7a Commissione sono state sollevate diverse eccezioni, relativamente alle competenze attribuite al Ministro dell'istruzione, università e ricerca dal comma 2, lettere *a)* e *c),* dell'articolo 1, ritenuto lesivo dell'autonomia universitaria, ai sensi dell'ordinamento vigente. Il testo approvato dalla Camera dei deputati è di fatto anteriore alla riforma dell'università (legge n. 240 del 2010). Secondo il mio modesto parere il citato comma 2, non incide in maniera estremamente negativa sulla legge n. 240. Si rammenta, al riguardo, che la nozione di crediti formativi universitari è stata introdotta dall'articolo 5 del decreto ministeriale del 1999, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei (poi sostituito, ma non modificato per questa parte); essi misurano l'impegno complessivo richiesto allo studente, comprensivo dello studio individuale, ma anche della partecipazione alle lezioni, alle esercitazioni, a tirocini e ad attività di orientamento. A ciascun credito corrispondono di norma 25 ore di lavoro. Il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti. Per conseguire la laurea occorrono 180 crediti; per la laurea magistrale, ne occorrono 120. La legge n. 240 del 2010, all'articolo 14, modifica l'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, riconoscendo che le università possono disciplinare nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a dodici. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Concordo con le esplicitazioni della collega Mariapia Garavaglia, riguardo «la promozione del merito che non si riscontra solo nel raggiungimento dei risultati, bensì anche nella valorizzazione del contenuto proprio di ciascuna disciplina». In ogni caso, si può ritenere che il comma 2 non stravolga la disciplina in vigore risultando addirittura ultroneo, in quanto si pone nell'ottica di favorire il riconoscimento dei crediti. L'auspicata approvazione del provvedimento nella versione originaria dell'abrogazione secca dell'articolo l-*septies*, volta a rispettare l'autonomia universitaria, avrebbe posticipato a lungo l'approvazione di un provvedimento, il cui scopo principale è di ripristinare è di ripristinare un criterio di ragionevolezza, considerata la particolare delicatezza della figura sanitaria professionale del fisioterapista, in quanto dedicata a compiere una funzione particolarmente importante nella riabilitazione dei pazienti.

io alla Camera definii quella norma clientelare ed elettorale - scelse di favorire l'illusione di tanti giovani laureati in scienze motorie, i cui posti di lavoro venivano sistematicamente tagliati nel mondo della scuola, di avere un percorso agevolato, o meglio, addirittura, l'equipollenza con la laurea in fisioterapia. Continuavamo, infatti, ad essere gli ultimi in Europa per ore di educazione fisica o di attività sportiva nella scuola e contemporaneamente si favorivano promesse illusorie, anche se la Camera nella stessa seduta, raggiungendo il massimo dell'ipocrisia politica, approvava un ordine del giorno della stessa maggioranza che impegnava il Governo a modificare un provvedimento non ancora approvato e pubblicato. Durante la XV legislatura si tentò, su iniziativa soprattutto del sottosegretario Dalla Chiesa, di arrivare ad una abrogazione semplice del provvedimento, ma la fine anticipata della legislatura impedì la conclusione del In questa legislatura il Senato aveva già approvato, con voto unanime in Commissione, l'abrogazione *sic et simpliciter* dell'equipollenza,

che in pratica si affida una nuova delega al Governo, che già deve predisporre numerosi regolamenti per la nuova legge sull'università. Allora permettetemi - colleghi, vi chiederei maggiore attenzione - qualche considerazione. L'approvazione dei colleghi della Camera ha preceduto la nuova legge n. 240 del 2010 sull'università, ovvero non vi era l'impegno del Governo ad approvare tutta una serie di provvedimenti riguardanti l'università. Ne aggiungiamo un altro entro nove mesi? Questo ulteriore provvedimento lede l'autonomia universitaria sui crediti, che erano già limitati dalla stessa legge sull'università.

I Capigruppo di maggioranza hanno poi ritirato la firma per evitare un nuovo passaggio alla Camera. Ma chiedo e vi chiedo: perché illudere nuovi giovani laureati? Perché non fare proposte serie a questi giovani nel mondo della scuola? Perché non tener presente che gli accessi alle facoltà di fisioterapia nelle università sono a numero chiuso e questo creerà ulteriore confusione alle stesse università, anzi falserà le ulteriori nuove ammissioni? Perché da parte di autorevolissimi Capigruppo della maggioranza in Commissione è stata ritirata la firma a questo emendamento, magari auspicando o suggerendo che il Governo non faccia in tempo a presentare poi il decreto?

ci ha detto il vice ministro all'istruzione Pizza? Forse sono solo alcune considerazioni illogiche, che però mi sento di proporre all'Aula. Il giorno dopo l'approvazione di questo provvedimento, quei giovani laureati in scienze motorie chiederanno giustamente l'attuazione della norma. Facciamo loro, come Parlamento, come Senato, proposte serie nel mondo della scuola e nel mondo dello sport. Non offriamo solo false illusioni. Approviamo tutti insieme un provvedimento votando l'unico emendamento presentato, che in Commissione era stato sottoscritto da tutti i Capigruppo presenti. di un gesto di serietà e - aggiungo e concludo - oltre tutto di coerenza verso la legge sull'università che avete da poco approvato. signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi,

che equiparò il diploma di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia, attribuendo lo stesso valore legale a titoli di studio conseguiti in base a percorsi formativi assai diversi. Mentre infatti per il conseguimento del diploma di laurea in fisioterapia è previsto un esame finale con valore abilitante alla professione sanitaria, tutto ciò non è contemplato per il corso di laurea in scienze motorie. Inoltre, tale equiparazione è in palese contrasto sia con le norme comunitarie in ordine alla formazione dei professionisti sanitari, sia con l'articolo 5 della legge n. 43 del 2006 sull'individuazione di nuove professioni in ambito sanitario. Né va inoltre dimenticato che lo stesso articolo 2, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 1998, istitutivo del corso di laurea, esclude per i laureati in scienze motorie la possibilità di svolgere attività di tipo sanitario. Va anzi ricordato che, già all'atto dell'approvazione del decreto-legge n. 250, alla Camera dei deputati fu accolto un ordine del giorno che impegnava il Governo a risolvere l'anomalia determinatasi a seguito dell'equipollenza tra i due diplomi di laurea. Nella legislatura successiva - la XV - furono immediatamente presentati, sia alla Camera che al Senato, disegni di legge volti ad abrogare l'articolo in questione. Alla Camera, dove ebbe inizio l'esame del provvedimento, ben presto emerse l'esigenza di trovare una mediazione con le aspettative dei laureati in scienze motorie. motorie. Alla fine, fu approvato un testo che demandava ad un decreto del Ministro dell'università la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi e delle modalità di espletamento di corsi di formazione e tirocinio ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia da parte dei laureati in scienze motorie. Quando il testo pervenne all'esame del Senato, la tendenza prevalente fu quella di limitare la portata dell'intervento alla sola abrogazione dell'equipollenza, in considerazione dell'effettiva difformità fra i due corsi di laurea; tuttavia, in un'ottica di mediazione rispetto alla scelta compiuta dall'altro ramo del Parlamento, fu convenuto di mantenere aperta la possibilità di conseguire il diverso diploma di laurea imponendo peraltro il rispetto della normativa vigente. La scelta perciò di rendere incompatibile con la professione sanitaria fisioterapica il laureato in scienze motorie è dettata dall'esigenza di dover tutelare gli ambiti professionali propri del fisioterapista, ma vuole al contempo richiamare il legislatore, magari tramite successivo intervento normativo, all'esame delle importantissime problematiche inerenti gli sbocchi occupazionali per il laureato in scienze motorie, al quale - tramite il ricorso ad uno stratagemma legislativo, quale l'emendamento di un decreto-legge estraneo per materia - si è riservata un'aggiunta che non risolve, anzi aggrava, l'assenza di una apposita professionalità del settore. A cosa mira allora il presente disegno di legge? Esso tende a riconoscere che soltanto il laureato in fisioterapia sia laureato di area sanitaria ed in quanto tale sia autorizzato - attraverso l'intervento e le manovre terapeutiche - a riabilitare la funzionalità di strutture fisiche colpite da forme patologiche, mentre al laureato in scienze motorie è riservato il compito di "adattare" le funzioni motorio-sportive alle condizioni del soggetto senza pretese di carattere terapeutico-riabilitativo, così come peraltro sottoscritto tra le associazioni delle diverse categorie nella cosiddetta Carta di Udine. Da qui, le conclusioni maturate in questa nuova lettura del disegno di legge afferente l'abrogazione dell'articolo 1, dove il Senato era e resta contrario a qualunque forma di *ope legis* o di modifica settoriale della normativa di carattere generale a vantaggio di determinate categorie. Nell'attuale legislatura il testo del disegno di legge, oggi al vaglio dell'Assemblea, è stato presentato nella versione originaria dell'abrogazione secca dell'articolo 1-*septies.* In tal senso, si è resa pertanto necessaria una nuova forma di mediazione, simile peraltro al testo licenziato dal Senato nella XV legislatura; nel senso che è confermata la consonanza del Ministero della salute sul decreto attuativo dell'università e, soprattutto, viene confermata la selezione per l'accesso. Si rende necessario e indispensabile compiere ora una scelta definitiva tra abrogazione secca e configurazione di un percorso per il passaggio dall'uno all'altro diploma di laurea. A tutto ciò si aggiunga che, durante questo percorso, l'*iter* del provvedimento non è stato privo di alcuni passaggi piuttosto travagliati e confusi, tra cui trasferimenti alla sede legislativa dapprima concessi, poi ritrattati. In questa scelta difficoltosa, tuttavia, la Commissione non ha fatto mancare il proprio sostegno con il senso di responsabilità che ne ha finora ispirato il comportamento. Tutti quanti abbiamo ben presente le difficoltà di sbocchi professionali che incontrano i laureati in scienze motorie, tanto da aver previsto per loro, con il disegno di legge n. 796 del 2008, un diverso percorso. C'è da dire, inoltre, che il provvedimento è stato presentato anteriormente alla legge n. 240 del 2010 di riforma dell'università, la quale ha un'impostazione alquanto rigorosa. Per cui, ci siamo interrogati sulla possibilità o meno di disciplinare a livello nazionale il riconoscimento dei crediti - che attualmente rientra nell'autonomia universitaria - ipotizzando la eventuale definizione soltanto di criteri generali. In ogni caso, è stata convinzione unanime che la strada dell'equipollenza dei relativi titoli di studio non era affatto percorribile e che ciò avrebbe comportato gravi conseguenze ai danni della salute dei cittadini. Non solo. Ma a ciò si aggiunga, inoltre, che il corso di laurea in scienze motorie non è aderente al profilo professionale dei fisioterapisti, né al *curriculum* europeo. Essa, cioè, renderebbe inefficace la programmazione annuale nazionale per l'accesso alla laurea in Fisioterapia, la cui impostazione viene disposta - com'è noto - sulla base di dati regionali. Altro fattore importante è il fatto che l'equipollenza non determina l'automatica abilitazione all'esercizio della professione di fisioterapista, ma essa, com'è noto, si consegue piuttosto superando l'esame di laurea in fisioterapia avente valore abilitante. Non v'è dubbio, allora, che la centralità dello snodo, vale a dire il punto essenziale del disegno di legge, è rappresentato dal comma 1, inerente l'abrogazione, mentre i commi 2 e 3 non stravolgono assolutamente la disciplina in vigore. La scelta, allora, è fra l'abrogazione secca dell'equipollenza e la mediazione raggiunta nella scorsa legislatura, tra Camera e Senato, fermo restando che la normativa vigente già affida alle università il compito di definire, nella loro autonomia, la disciplina del riconoscimento dei crediti. Ho avuto modo, a suo tempo, di manifestare le mie perplessità, quando fu approvato l'articolo 1-*septies*. Oggi, però, alla luce dell'articolato dibattito sviluppatosi nei due rami del Parlamento e della piena disponibilità ad individuare modalità idonee ad una rapida approvazione,

si tratta di due lauree importanti, senza alcun dubbio. È la valorizzazione della dignità delle professioni scelte che fa sì che noi dobbiamo valorizzarle entrambe. Non è possibile dover consentire una via di uscita laterale per chi, avendo scelto una professione, essendo rimasto senza insegnamenti ed occupazione, ha bisogno che ci sia una equipollenza: per fare cosa, Ministro, Sottosegretario, colleghi? Per accedere alla preparazione ad una professione di carattere sanitario. Badate bene che la fisioterapia è essenziale nella riabilitazione e, stante le tante e diverse cure di lungo periodo e di alta qualificazione, c'è bisogno addirittura del fisioterapista con specializzazioni. Come facciamo ad ottenere la specializzazione di un professore di educazione fisica? Di questi, hanno bisogno i giovani. Il Ministro della pubblica istruzione piuttosto aumenti le ore di scienze motorie. Là abbiamo la prevenzione di scoliosi e obesità,

né dei laureati in scienze motorie. Perciò chiederei all'Assemblea una attenzione molto particolare. È un provvedimento che sembra piccolo perché di breve discussione, ma è di grande importanza rispetto al destino di coloro che hanno raggiunto queste lauree lauree e dei titolari del diritto alla tutela della salute. Inoltre, Presidente e colleghi, nel 2010 abbiamo approvato la legge n. 240 sul riordino dell'università. Addirittura si possono accorpare o abolire facoltà. Il Ministro chiede la riduzione dei corsi di laurea: qui abbiamo a che fare con una laurea a a numero programmato, come tutte le altre professioni in sanità, ma ora introduciamo un elemento di disturbo grave anche dell'autonomia universitaria. Viene compiuta nuovamente una scelta centralista, che va contro gli interessi di tutti: di coloro che scelgono una laurea, dei cittadini italiani che hanno bisogno di servizi diversificati di prevenzione e di riabilitazione, e anche del Ministero dell'istruzione, dell'università

l'emendamento 1.100, unico emendamento presentato in Assemblea sul provvedimento in esame, rappresenta, come già ampiamente detto nel mio precedente intervento in discussione generale,

della Commissione in sede legislativa - le condizioni politiche sono mutate. L'Italia dei Valori vuole rispettare appieno l'impianto legislativo approvato dalla Camera dei deputati dei deputati e, pur avendo presentato lo stesso emendamento in Commissione, non potrà votare favorevolmente sullo stesso solo ed esclusivamente per evitare il pericolo di un ennesimo rimpallo di questo provvedimento

Presidente, anch'io sono dispiaciuto del rapporto tra maggioranza e opposizione in quest'Aula.

al comma 1 dell'articolo 1, non riesco a comprenderlo. Per questo motivo voteremo contro l'emendamento 1.100 in modo da porre termine a una questione che ormai da troppo tempo si dibatte nel Paese e finalmente trova la giusta soluzione.

voterà senz'altro a favore di questo provvedimento, che deve essere approvato nel più breve tempo possibile.

Invito tutti i colleghi intervenuti, soprattutto quelli che fanno parte della 7a Commissione e hanno presentato questo emendamento, a rileggersi i propri interventi in quella

la legge sull'università. Penso che un po' di coerenza ognuno di noi dovrebbe mantenerla, e il Gruppo del Partito Democratico in Commissione e in Aula decide di farlo. Ci vorrebbe un quarto d'ora: ne abbiamo parlato anche con i colleghi alla Camera (perché noi ci parliamo con i colleghi della Camera). Voglio ricordare un dato che ho citato prima in discussione generale: quando la Camera ha approvato questo provvedimento non vi era ancora la nuova legge sull'università, la n. 240 del 2010: vorrei che ciò rimanesse agli atti. Per

Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, colleghi, credo che, dopo oltre cinque anni di vigenza di questa norma, sia giunto il momento di rimediare a questo grande errore. Credo che in passato, e anche qui oggi, si sia già detto tutto su questa annosa vicenda: ogni Gruppo e ognuno di noi ha potuto acclarare i propri convincimenti. Pur non condividendo le tesi di tutti, e soprattutto senza tornare sulle motivazioni che spingono l'Italia dei Valori a votare a favore di questo provvedimento, ritengo di poter senza alcun dubbio affermare che le due professioni

Un'Aula così affollata, numerosa e disattenta è il massimo del massimo. Quindi, chi resta qui o ascolta il senatore Caforio, o tace, oppure, se vuole chiacchierare, aiuta tutti uscendo fuori Veramente difficile seguire i lavori dell'Aula Mi riferisco all'errore madornale che molte facoltà di medicina hanno fatto quando, per vari motivi e - perché no - interessi, hanno deciso di ospitare corsi di laurea in scienze motorie. Questa è stata la decisione che ha creato false aspettative ed illusioni. Il tutto poi, in presenza di un altissimo tasso di disoccupazione per una categoria e di una quasi totale occupazione per l'altra, ha accentuato il fenomeno dell'abusivismo, tenuto conto anche del fatto che questo Parlamento ancora non è stato e non è in grado di completare il ciclo di riforma delle allora «arti sanitarie». Ciclo di riforma che prevede l'istituzione di ben 22 profili professionali, dei relativi corsi di laurea e di altrettante professioni sanitarie (non mediche), nonché l'istituzione dei relativi ordini ed albi, regolamentando così questo delicatissimo settore. Per spiegare la mia perseveranza nel volere l'abrogazione della equipollenza tra i due titoli, permettetemi di toccare la mia sfera personale, e di ciò vi chiedo anticipatamente scusa. Sono anch'io un professionista sanitario. Sono laureato in tecnica ortopedica e, nel mio lungo percorso professionale e lavorativo (circa quarant'anni), ho lavorato spessissimo fianco a fianco con fisioterapisti: ho quindi avuto modo di apprezzare il loro lavoro, unico ed indispensabile nel recuperare e riabilitare pazienti affetti da gravi patologie dell'apparato locomotore. In sintesi, tanto per fare un esempio, colleghi e chiedo un minimo di attenzione dell'Assemblea, signor Presidente - io non farei mai manipolare la mia colonna vertebrale da un laureato in scienze motorie, pur bravo che possa essere, né tanto meno farei seguire un bambino cerebroleso allo stesso professionista. Sfido chiunque in quest'Aula a sostenere che, per curare la propria cervicale, preferirebbe un intervento dì un laureato in scienze motorie, così come è formato, alla luce delle norme in vigore e dei percorsi formativi attualmente attivati. per curare le patologie servono medici e professionisti del settore sanitario. I laureati in scienze motorie che vorranno cimentarsi in questo delicatissimo settore potranno sempre e comunque farlo dopo aver acquisito con lo studio e con la pratica non *ope legis* - tutte le competenze già previste dall'ordinamento universitario. Per questo, Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori all'Atto Senato n.

Mi sembra che fu in un contesto profondamente sbagliato che si volle dare una risposta a tutti i costi ad una categoria che già soffriva della scarsa possibilità di occupazione. Si fece una cosa sbagliata perché si equiparò quello che non si poteva equiparare, forse sulla scorta di qualche idea insana secondo la quale alcuni esami che avevano lo stesso nome potevano far pensare che poi si avesse il titolo per fare la stessa professione, con qualche modesto correttivo. Sono certo che colleghi avvocati sappiano molto di medicina legale, ma non potrebbero mai fare un'autopsia; viceversa, dei medici specialisti in medicina legale non potrebbero affrontare da avvocati un processo.

altrettanto sbagliato nel voler disciplinare a tutti i costi l'accesso a una facoltà a numero chiuso per studenti che hanno conseguito un altro tipo di titolo

dobbiamo deglutirne un'altra che ne ha meno e che palesemente confligge, come è stato perfino detto dal relatore, con l'attuale normativa che disciplina l'università. Lo facciamo volentieri sapendo di far cosa migliore rispetto a quella di lasciare le cose così come sono. Fa molto pensare il dover agire per forme costrittive piuttosto che per libere scelte; fa molto pensare anche sul nostro stesso ruolo, ma tant'è. Votiamo quindi a favore di questo provvedimento, convinti che possa far meglio che peggio. *(Applausi Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il disegno di legge in esame è volto ad abrogare l'articolo che ha disposto l'equipollenza della laurea in scienze motorie alla laurea in fisioterapia, subordinatamente alla frequenza certificata di un «corso su paziente» da istituire presso le università con un decreto ministeriale. Il provvedimento era stato già esaminato nel corso delle due precedenti legislature sia dalla Camera che dal Senato, giungendo all'approvazione di un testo che teneva conto dell'esigenza di salvaguardare gli iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie che, nelle more dell'adozione della disciplina di coordinamento, si fossero iscritti o fossero già iscritti al corso di laurea in scienze motorie con l'aspettativa di un'equipollenza con quello di fisioterapia. Per questo motivo, il testo del progetto di legge approvato all'unanimità in sede legislativa dalla Commissione cultura della Camera, nel corso della XV legislatura, inseriva un nuovo comma 2 all'articolo in esame, ai sensi del quale si prevedeva che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, si definisse per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi, nonché delle modalità di espletamento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia. Le modifiche approvate dal Senato prevedevano che il decreto fosse adottato di concerto con il Ministro della salute; vi fosse la precisazione della necessità del rispetto della normativa vigente nella definizione del menzionato decreto; si trattasse poi di crediti formativi utili ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia; la necessità per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie di superare una prova di selezione per l'accesso ai posti complessivamente programmati in fisioterapia nei limiti del fabbisogno previsto. Le competenze professionali del fisioterapista sono quelle di attuare protocolli che prevedono un importante utilizzo di terapie manuali, come massaggi e mobilità passiva; sviluppare protocolli che necessitano dell'utilizzo di apparecchiature di energia fisica di tipo semplice e complesso in presenza della figura medica specialistica ovvero del fisiatra, quali laser, ultrasuoni, ionoforesi. Al contrario, le competenze professionali del laureato in scienze motorie sono quelle di attuare protocolli di adattamento fisiologico attraverso la prescrizione e la pratica di esercizi di mobilità attiva, anche per categorie quali cardiopatici, diabetici, obesi gravi; esercizi fatti svolgere anche con macchinari volti agli adattamenti muscolari, come macchine isotoniche, isocinetiche, e con macchinari volti all'allenamento cardiovascolare. Si tratta, quindi, di protocolli di attività che possono essere svolti secondo modalità attiva o passiva, a seconda dei casi e delle situazioni e che comunque non richiedono un diretto contatto manuale tra terapista e paziente; protocolli di valutazione e rieducazione degli schemi motori e delle capacità motorie come propriocezione, ginnastica posturale e adattiva. Vi sono quindi forti analogie tra i due corsi di laurea, sebbene riteniamo importante che chi intende chiedere il riconoscimento dei crediti per l'accesso al corso di laurea in fisioterapia debba necessariamente svolgere il tirocinio secondo le modalità di quel corso di laurea, altrimenti potrebbero ingenerarsi incertezze interpretative sul tipo di formazione e tirocinio sul paziente da far eseguire da parte del laureato in scienze motorie che voglia accedere al corso di laurea in fisioterapia. In sede di discussione nella sede referente è emersa, in prima istanza, la necessità di approvare il provvedimento nella versione originaria dell'abrogazione secca dell'articolo l-*septies*, volta a rispettare l'autonomia universitaria. Il testo approvato dalla Camera dei deputati è di fatto anteriore alla riforma dell'università (legge n. 240 del 2010), che prevede il riconoscimento di dodici crediti, sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente, escludendo forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Ci associamo all'invito rivolto dal Governo a procedere all'approvazione del disegno di legge in titolo, anche al fine di contribuire ad elevare il livello effettivo di tutela della salute, nel rispetto e nella valorizzazione delle competenze di tutti i soggetti coinvolti, a cominciare dalle Regioni.

perché finalmente si raggiunge l'obiettivo di abrogare l'articolo 1-*septies* del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Ma oltre questa considerazione rimane la delega al Governo per un nuovo provvedimento, entro i prossimi nove mesi, per l'accesso dei laureati in scienze motorie alle facoltà di fisioterapia, di cui non avvertivamo alcuna necessità, che produrrà inutili illusioni in giovani laureati che invece avrebbero diritto a posti di lavoro veri nella scuola italiana, la più povera di attività fisiche e sportive in Europa; che susciterà confusione per l'accesso alle facoltà a numero chiuso di fisioterapia; che viola, di fatto, l'autonomia universitaria e il relativo riconoscimento dei crediti. Migliaia di giovani aspettavano progetti e proposte serie per realizzarsi professionalmente. Per fare questo occorreva non tagliare risorse sulla scuola, come invece è stato fatto sistematicamente in questi tre anni. Auspico che il Governo non pensi di rispondere a queste giuste attese con inutili illusioni. Nonostante questo, confermiamo il voto favorevole, perché finalmente viene abrogata la norma iniqua del febbraio 2006. *(PdL)*. Signor Presidente, siamo qui oggi per discutere un provvedimento che credo non sarà difficile approvare, anche con la collaborazione dei colleghi dell'opposizione. mi auguro che così possa accadere. Mi preme però fare una piccola premessa, che credo possa essere altrettanto condivisa dai colleghi e che, anche se affronta il problema da una via, per così dire, laterale, vale certamente la pena discutere. Anche nella Commissione di cui sono componente - la 7a Commissione - e in cui si è affrontato questo disegno di legge, è emerso che non è certamente semplice conciliare i piani di riforma del Governo e del Parlamento senza andare ad intaccare la giusta autonomia che ogni ateneo ha il diritto di rivendicare; libertà d'azione che, correttamente, viene comunque riconosciuta ad ogni singolo ateneo del Paese. Eppure, proprio questa tanto rivendicata autonomia ha rischiato da anni di mettere in crisi lo stesso sistema universitario; in particolar modo per quanto concerne la straordinaria proliferazione di corsi e corsi di studio, creati ad arte più per interessi particolari che non nel preciso interesse degli studenti italiani. Un aumento esponenziale di corsi e facoltà che spesso si sovrappongono l'uno sull'altro, creando un'incredibile confusione e un senso di spaesamento negli stessi studenti. Creare dei corsi di studio al fine di offrire una preparazione meno generalista per i nostri ragazzi era uno scopo utile anche per creare professionalità maggiormente specializzate e più qualificate per il mondo del lavoro; era un modo per "modernizzare" il nostro sistema universitario, troppo spesso molto preoccupato di offrire un'ottima cultura generale ai propri allievi, ma uno scarso profilo specialistico e soprattutto pratico. In troppe occasioni però ciò ha significato - purtroppo spesso - la creazione di corsi di studio obsoleti e inutili, difficilmente spendibili dai nostri studenti presso le aziende e le società. Oggi la nostra preoccupazione è proprio quella di cercare di rendere quanto più efficace possibile la relazione tra il sistema economico e il sistema universitario del nostro Paese. Credo che la recente approvazione della riforma universitaria da parte delle Camere, nello scorso dicembre, possa essere una buona base da cui partire per permettere un più proficuo dialogo tra laureati e mondo del lavoro; ma molto bisogna ancora fare e, soprattutto, c'è bisogno di una costante collaborazione proprio dai diversi atenei italiani, che non possono arroccarsi, ma devono confrontarsi con equilibrio ed aprire un dialogo produttivo anche con la politica, nel preciso interesse degli studenti e del loro futuro. e fatta questa doverosa premessa, possiamo prendere in esame da una più ampia prospettiva il provvedimento all'ordine del giorno. L'equipollenza tra due titoli di studio quali scienze motorie e fisioterapia può sicuramente apparire come una sorta di nonsenso: sono due corsi che hanno in comune alcune materie di studio, ma che solo apparentemente possono sembrare uguali, nonostante si orientino in un certo qual modo nella stessa branca scientifica. Eppure sono due corsi diversi fra loro e, soprattutto, con differenti obiettivi: uno - quello di scienze motorie può avere finalità di prevenzione medica; l'altro - quello di fisioterapia - ha scopi curativi e riabilitativi. Non è quindi possibile rendere uguali due corsi con così differenti applicazioni. Inoltre, come segnalatomi da diversi studenti, se convalidassimo una secca e automatica equipollenza tra i due diplomi di laurea, avremmo commesso una vera ingiustizia nei confronti dei laureati in fisioterapia che, per accedere a questi particolari corsi, hanno dovuto superare un test d'ingresso con pochissimi posti disponibili: questi studenti hanno quindi dovuto superare già in partenza una selezione molto stringente. L'accesso ai corsi di scienze motorie è invece soltanto a volte a numero chiuso, ma con una disponibilità di posti ampiamente maggiore rispetto a quelli di fisioterapia. I laureati in fisioterapia inoltre, per i motivi appena citati, hanno in genere anche maggiori possibilità di inserirsi più rapidamente nel mondo del lavoro, ma oggi commetteremmo comunque un errore, se non ci interessassimo dei problemi degli sbocchi lavorativi per i laureati in scienze motorie. Bisognerà discutere e quindi approvare al più presto il disegno di legge (Atto Senato n. 796) sull'accesso professionale dei laureati in scienze motorie, in modo tale che, con l'abrogazione dell'equipollenza con il diploma di laurea in fisioterapia, non si finisca per favorire degli studenti e svantaggiarne poi altri. Non possiamo assolutamente permetterci di lasciare abbandonati a sé stessi i laureati in scienze motorie. L'Atto Senato n. 796 si propone specificamente che nelle palestre e nelle strutture sportive debba essere obbligatoria la direzione di un laureato in scienze motorie: ciò renderebbe giustizia agli anni di studio compiuti da questi ragazzi e garantirebbe loro di mettere al servizio della comunità le proprie abilità. In Italia ci sono circa sei milioni di persone che praticano un'attività sportiva, spesso senza alcuna tutela preventiva circa gli esercizi che dovrebbero svolgere in base alle proprie esigenze fisiche. Sarebbe quindi utilissimo poter offrire a tanti sportivi l'assistenza di un preparatore o di un allenatore esperto e capace, facendo leva proprio sul percorso di studi svolto. Per concludere, resto quindi favorevole all'abrogazione dell'equipollenza tra i due corsi di studio presi in esame quest'oggi, ma ritengo altresì che debbano essere messi in campo tutti gli sforzi da parte delle Camere e del Governo per avviare al più presto un'efficace discussione sugli sbocchi professionali dei laureati in scienze motorie, secondo un'opinione già condivisa da gran parte della Commissione istruzione pubblica e beni culturali, e che credo troverà una sollecita risposta da parte del Governo. In gioco c'è il futuro di tanti ragazzi, che reclamano giustizia e garanzie per poter più serenamente pianificare il proprio avvenire. Abbiamo il preciso dovere di mettere in campo tutte le nostre energie affinché ciò possa accadere. È per questi motivi che dichiaro il voto favorevole del PdL a questo provvedimento. La ringrazio, signor Presidente.

parlamentare Lo Presti e altri sulla modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. Il relatore, senatore Zanoletti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'11 maggio 2010 la Camera dei deputati ha approvato, con 499 voti favorevoli e uno solo contrario, il disegno di legge di iniziativa parlamentare Lo Presti e altri sulla modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. Ricordo che le casse di previdenza, cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali, sono state privatizzate dal 1° gennaio 1995, nell'ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, di 15 enti. Gli enti, una volta privatizzati, hanno continuato a sussistere come enti senza scopo di lucro, assumendo la personalità giuridica di diritto privato (ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile) e subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali. Successivamente, la legge 8 agosto 1995, n. 335 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare") ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In attuazione di tale norma è stato emanato il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha assicurato a decorrere dal 1° gennaio 1996 la tutela previdenziale per i richiamati soggetti. In attuazione di tale decreto sono stati istituiti 5 enti privatizzati. Ai sensi dell'articolo 2 del medesimo le associazioni o fondazioni hanno autonomia gestionale organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti e in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta. In particolare, l'articolo 2 ha disposto l'applicazione per tali enti del sistema del calcolo contributivo. Inoltre, gli iscritti alle casse professionali sono tenuti, in virtù dei singoli regolamenti di gestione, al versamento di specifici contributi. Tali regolamenti stabiliscono, in primo luogo, la misura del contributo soggettivo legato principalmente al reddito dell'iscritto, luogo, la misura del volume di affari annuale su cui calcolare un contributo integrativo del 2 per cento. La situazione venutasi a creare ha portato ad erogazioni molto basse per i più di 200.000 iscritti. Pensioni basse dovute sia alla ridotta quota dei contributi soggettivi (solo il 10 per cento), sia ai bassi redditi dichiarati, sia alla limitata storia contributiva. La norma approvata dalla Camera propone, per il contributo integrativo, invece della misura fissa pari al 2 per cento del fatturato lordo, una misura stabilita con delibera dell'ente cassa dell'ente cassa competente, approvata dai Ministeri vigilanti, fermo restando che il contributo integrativo sia determinato in percentuale del fatturato lordo. In ogni caso, la delibera non può prevedere una aliquota superiore al 5 per cento. Il contributo integrativo, come prevede anche la norma vigente, è riscosso dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento del corrispettivo da parte del cliente, previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura. La legge approvata dalla Camera concerne, oltre ai regimi pensionistici di cui al citato decreto legislativo n. 103, anche quelli di istituzione antecedente e che abbiano adottato o adottino il sistema di calcolo contributivo. Inoltre, la novella in oggetto prevede che, per i regimi summenzionati, l'ente cassa competente possa destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali dei contributi al fine di migliorare i trattamenti pensionistici. La delibera di tali enti è adottata secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente nonché dallo statuto e dal regolamento dell'ente o cassa ed è approvata dai Ministeri vigilanti.

La Commissione lavoro del Senato ha ritenuto, all'unanimità, opportune le modifiche contenute nel testo della Camera, dichiarandosi anche disponibile a chiedere l'assegnazione in sede deliberante. È evidente, infatti, che in tal modo è possibile incrementare i montanti contributivi assicurando pensioni più decorose e dando una prospettiva di maggior tranquillità ai giovani professionisti. Per essi le previsioni, allo stato, sono un tasso di sostituzione anche inferiore al 30 per cento, e dunque assolutamente insufficiente. Le categorie interessate hanno manifestato in varie forme il loro favore e la loro aspettativa per una rapida conclusione dell'*iter* legislativo. Le Commissioni competenti del Senato in sede consultiva hanno espresso parere favorevole; anche il Governo si è pronunciato in tal senso.

Si tratta - come è evidente - di modifiche non sostanziali che la Commissione lavoro ha fatto proprie, approvando sempre all'unanimità un emendamento del relatore, ed è in questa forma che il testo giunge all'esame dell'Aula. Confido in una rapida approvazione, perché è un passo limitato ma significativo sul percorso del necessario adeguamento delle norme pensionistiche alla mutata realtà sociale e finanziaria.

nel corso del suo *iter* questo disegno di legge aveva incontrato alla Camera la sostanziale unanimità dei Gruppi. Anche nella Commissione lavoro al Senato l'accordo è stato generale e se ne era richiesta addirittura - come ha detto il relatore - l'assegnazione in sede deliberante. Il sistema previdenziale dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione presenta una struttura peculiare, assai differente rispetto a quello previsto per il lavoro dipendente, per quanto concerne gli organismi deputati a garantire quei «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» cui, in base all' articolo 38 della Costituzione, tutti i lavoratori hanno diritto. Il settore vanta un'esperienza ormai quindicennale per le casse «storiche» (quelle privatizzate in base al decreto legislativo n. 509 del 1994) e ormai ultradecennale per quelle «di seconda generazione» (costituite con il decreto legislativo n. 103 del 1996). Si tratta di una esperienza la cui valutazione complessiva è senza dubbio positiva, sebbene la necessità di interventi correttivi del legislatore sia davvero necessaria. I liberi professionisti, al pari dei lavoratori dipendenti, hanno diritto a beneficiare di adeguate prestazioni previdenziali e assicurative, cosa che attualmente non avviene in quanto essi percepiscono pensioni significativamente basse con una grossa disparità rispetto al reddito percepito nel corso dell'attività professionale. Mi si consenta qui di ricordare come sia particolarmente grave la situazione delle professioniste donne. Secondo le statistiche, infatti, esse percepiscono una pensione che ammonta a circa la metà di quella degli uomini, scontando inoltre i periodi di interruzione dovuti alla maternità e ai servizi di cura della famiglia. Una situazione che ricalca purtroppo quella che caratterizza il settore del lavoro dipendente, dove le donne risultano essere particolarmente penalizzate. La possibilità di aumento delle aliquote è uno strumento per tentare di sanare almeno in parte una situazione di disparità di trattamento estremamente sfavorevole per alcune casse previdenziali. Esiste, inoltre, un concreto pericolo per questi enti, soprattutto se di recente istituzione. Molti di essi, infatti, si trovano oggi in una situazione apparentemente invidiabile dal punto di vista delle risorse finanziarie, poiché ad un buon numero di professionisti contribuenti si affianca un numero relativamente basso di pensionati utenti. Il rischio ovvio è che, proseguendo nella gestione, si possa registrare un significativo peggioramento dei bilanci, nel momento in cui la tendenza cominciasse anche solo a riequilibrarsi e tali casse dovranno cominciare ad erogare un numero significativo di prestazioni. In seguito all'adozione, da parte delle casse previdenziali privatizzate, del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche e della presenza di aliquote contributive estremamente contenute, in essere interventi volti ad incrementare la base di calcolo del trattamento pensionistico espressa dai montanti contributivi, in modo tale da garantire l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici in continuità con il reddito professionale

pur, forse, inevitabile. L'aumento dell'aliquota viene infatti riscosso direttamente dal professionista all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura: il cliente ha il diritto di essere informato, ma comunque pagherà questo aumento. D'altra parte il professionista, che vorrà accumulare una pensione più consistente, avrà tutto l'interesse a fatturare interamente i propri introiti e naturalmente questo sarà un miglioramento anche per il fisco. In conclusione, ribadisco qui quanto ho già sostenuto in Commissione lavoro: la proposta in discussione rappresenta senz'altro, a mio giudizio, un passo avanti compiuto in direzione di un sostegno concreto agli iscritti alle casse professionali. Da qui nasce l'adesione mia e del mio Gruppo.

della legge finanziaria del 2007 che, modificando l'articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, ha recato disposizioni per garantire l'equilibrio finanziario degli enti previdenziali che sono stati privatizzati. Questo non ha alcun impatto inflattivo, perché le prestazioni rese dai professionisti iscritti agli enti di previdenza privati, istituiti nel 1996, non sono inserite nell'elenco preso in evidenza dall'ISTAT, il famoso "paniere", ai fini del calcolo del tasso di inflazione. La misura del contributo integrativo non può eccedere il 5 per cento dal 2 per cento attualmente fissato. Voglio ricordare che abbiamo a che fare con un settore della previdenza obbligatoria che riguarda le casse privatizzate, una ventina di cui una parte - se ben ricordate - istituite con la cosiddetta riforma Dini del 1995. Ma cosa fa questa legge? Si propone di allineare le casse nuove, quelle riferite alla riforma Dini del 1995 e quelle del decreto legislativo n. 103 del 1996, per quanto riguarda il contributo integrativo, al tetto del 5 per cento delle altre casse. Queste ultime, le vecchie casse, non vedono stravolgimenti in quanto il contributo del 4 per cento o del 5 per cento già lo riscuotono. Quindi questo contributo viene destinato a prestazioni assistenziali e, se poi il disegno di legge verrà approvato, una parte di questo contributo potrà essere destinata a prestazioni previdenziali. Ricordo ancora che per le nuove casse si fa semplicemente un'operazione di allineamento alla situazione delle altre. Signora Presidente, il provvedimento che discutiamo oggi ha il compito di affrontare uno dei temi portanti della struttura del nostro *welfare*: quello della adeguatezza e della sostenibilità dei trattamenti pensionistici. Lo fa con riferimento a una categoria definita e limitata, quella degli esercenti le libere professioni, iscritti ad albi ed ordini professionali, titolari - come ha evidenziato il relatore

conseguente incertezza dell'orizzonte previsionale, l'andamento della gestione di queste casse ha risentito e risente della variazione nel tempo della dinamica demografica degli iscritti e di quella reddituale, soprattutto dei professionisti più giovani. L'aumento progressivo della longevità dei beneficiari delle prestazioni a fronte della riduzione della consistenza dei versamenti dei nuovi iscritti pone seri problemi di sostenibilità gestionale delle casse per la prospettiva. Alcune di queste hanno avuto in passato, e presentano anche attualmente, problemi di equilibrio di bilancio, derivanti anche da politiche di gestione non sempre oculate e coerentemente finalizzate allo scopo costitutivo. Altre, quelle di più recente istituzione, godono,

e se non saranno gestite con la massima trasparenza ed oculatezza. Per questa ragione, l'intervento promosso dal provvedimento è opportuno, poiché rappresenta comunque un vantaggio, un passo verso l'autonomia delle casse e a sostegno dell'adempimento delle loro finalità costituzionali. Ma se la sostenibilità gestionale è l'ovvio presupposto del pieno esercizio funzionale, è la sostenibilità dei trattamenti previdenziali erogati la fonte di vera preoccupazione, ciò di cui dovrebbe primariamente occuparsi il Parlamento. La previsione, contenuta in questa norma, che riconosce la facoltà per le casse che adottano il sistema di calcolo contributivo di destinare una parte del contributo integrativo, che qui viene incrementato, ad aumentare la consistenza dei montanti individuali può aumentare in futuro i tassi di sostituzione, ma probabilmente non in misura sufficiente. Le nuove casse pagano già attualmente pensioni molto basse, che segnano uno scarto marcato rispetto ai redditi medi della vita attiva, attiva, produttiva dei loro aderenti. Questo scarto colpisce in misura particolare e inaccettabile le professioniste donne, che arrivano a percepire pensioni che ammontano a circa la metà di quella dei colleghi uomini, a causa dei periodi di interruzione contributiva dovuti alla maternità e e agli impegni di cura in favore dei figli e della famiglia. È quanto mai necessario, quindi, affrontare in maniera sistematica il problema della riforma del lavoro autonomo, considerandolo anche nella prospettiva di genere ed estendendo alle professioniste

Inoltre, i nuovi iscritti, i giovani, hanno di fronte a se una prospettiva anche peggiore: stime attuariali calcolano che le categorie a reddito più debole e discontinuo iscritte alle "nuove" casse (ad esempio, i biologi, gli psicologi, gli agronomi) riceveranno pensioni pari a circa il 25 per cento del loro reddito medio, mentre ai giovani avvocati ed ingegneri di oggi, iscritti alle casse privatizzate, spetterà una pensione pari a circa il 50 per cento del reddito medio attuale dei giovani iscritti, che oggi si aggira tra i 1.200 e 1.600 euro al mese. Se si considera, inoltre, che molti di questi giovani iscritti sono "forzati" della libera professione, la esercitano, cioè, non per scelta, ma perché costretti da un mercato e da un costume che hanno cancellato, di fatto, il lavoro dipendente dal novero dei rapporti di lavoro, ci si rende ben conto dell'assoluta necessità di assumere il tema della sostenibilità sociale per la prospettiva dei trattamenti previdenziali di coloro che oggi entrano nelle professioni. Abbiamo a che fare, ancora una volta, con un problema sostanziale per il futuro: quello della qualità del lavoro dei giovani, della loro autonomia, in definitiva quello della costruzione dei presupposti per un Paese meno diseguale. Mancano, evidentemente, la voglia, il coraggio, il respiro per affrontare ciò che sarebbe necessario: una riforma complessiva della previdenza, delle quote di contribuzione per tutte le professioni, degli strumenti di accompagnamento alle fasi della vita lavorativa in un mercato del lavoro di grande mutevolezza, degli strumenti di qualificazione e di "normalizzazione" del lavoro. Ma anche a voler essere minimalisti e a mantenere il profilo ristretto alla normativa previdenziale e al testo di questo provvedimento, è necessario affrontare almeno l'armonizzazione di quello che c'è, se non si vuole affrontare quello che manca. Non possiamo quindi non richiamare la necessità di affrontare al più presto il tema della totalizzazione contributiva, prevedendo la possibilità per tutte le categorie di lavoratori, dipendenti od autonomi, quale che sia il loro percorso assicurativo, di cumulare tutti i periodi assicurativi, di qualunque durata ed acceso presso qualsivoglia ente, finalizzandolo al conseguimento di un'unica pensione che capitalizzi ogni singolo versamento contributivo effettuato nel corso della vita, senza dispersioni e penalizzazioni. Così come deve essere superata l'incongruenza e l'iniquità prodotta da recenti norme. Una fra tutte l'introduzione dell'onerosità per la ricongiunzione contributiva presso l'INPS dei contributi dalle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative, che determinerà per moltissimi lavoratori riduzioni significative dei montanti pensionistici ed in alcuni casi la perdita del requisito di accesso alla pensione. Non è per parlar d'altro, ma affrontare il tema previdenziale significa farsi carico del complesso dei problemi che riguardano il futuro previdenziale e pensionistico delle giovani generazioni. Per tutto quanto detto, ben venga l'intervento previsto da questo provvedimento, con la consapevolezza che però esso è assolutamente parziale e limitato e rischia in termini di prospettiva di essere perfino iniquo se non verrà completato il quadro delle necessarie riforme. Ricordiamoci delle criticità che esso pone in luce anche quando discutiamo dei limiti, sempre più forti, che si vorrebbero imporre all'accesso dei giovani ad alcune professioni: chi sosterrà la pensione degli stagisti, dei praticanti a titolo gratuito degli studi legali, dei tirocinanti per periodi infiniti se continuiamo a porre barriere protezionistiche e corporative all'accesso alle professioni? C'è molto lavoro da fare, ma quest'Aula, signora Presidente, me lo consenta, continua ad essere riempita di contenuti minimi, non sapendo affrontare, per debolezza politica della maggioranza, le questioni di sostanza che riguardano il Paese. Il provvedimento che discutiamo oggi avrebbe potuto essere approvato dalla Commissione referente in sede deliberante, è stata fatta richiesta, con l'accordo di tutti i Gruppi e con il parere favorevole del Governo. Ci troviamo a discuterlo in Aula, seppure in termini condivisi, ed è forte il sospetto che ciò si debba alla necessità di riempire un calendario altrimenti vuoto. Accade sempre più spesso ed è inaccettabile: per rispetto del Parlamento, ma soprattutto per rispetto dei cittadini, che hanno diritto ad istituzioni efficienti e pienamente impegnate nell'affrontare e risolvere i loro problemi. chiediamo che possano essere discusse dall'Aula del Senato al più presto le molte proposte in materia di lavoro e previdenza che sono state presentate dal nostro Gruppo proprio con questo intento.

per il disegno di legge in titolo e il relativo emendamento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo». «La Commissione programmazione «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo osservando che il provvedimento inserisce un elemento di finanziamento del montante previdenziale che, difformemente dal sistema vigente, non ha propriamente natura contributiva, ma viene posto a carico della fiscalità generale. Esprime altresì parere di nulla osta sull'emendamento 1.100».

Signora Presidente,

molto al di sotto del reddito percepito nel corso dell'attività professionale. Infatti, il disegno di legge in esame reca disposizioni volte a permettere agli enti previdenziali istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 di elevare la misura del contributo integrativo. Tale proposta è volta a equiparare sotto questo aspetto la disciplina relativa a tali enti a quella vigente per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto n. 509 del 1994. Riteniamo quindi che tale provvedimento possa essere accolto come primo atto necessario alla soluzione di un problema reale; ma riteniamo altresì che insieme ad esso vadano affrontati il riordino degli enti previdenziali privatizzati (con un riassetto organico della disciplina, da perseguire attraverso uno specifico intervento legislativo) e, più in generale, la necessità di garantire nei prossimi anni una pensione dignitosa ai nostri giovani, soprattutto ai giovani professionisti, che spesso oggi hanno uno stipendio bassissimo, vivono di *stage* e in futuro non avranno una pensione. Come ricorderete, il Governo Prodi con il Protocollo sul *welfare* del 2007 intendeva, da un lato, sostenere il secondo pilastro su cui si basava la riforma pensionistica che introdusse il sistema contributivo contributivo e la previdenza complementare e, dall'altro, garantire un tasso di sostituzione del 60 per cento nel rapporto tra retribuzione e pensione. Per quanto concerne la previdenza complementare sarebbe opportuno avviare una verifica attenta su quanto la crisi economica degli ultimi anni abbia depotenziato tale strumento

Questa parte del Protocollo non fu mai attuata a causa della fine anticipata della legislatura, ma il tema resta drammaticamente attuale. Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo PD al provvedimento in esame e nel ricordare che il Partito Democratico, come diceva la collega Ghedini, ha presentato molti disegni di legge sul tema del lavoro, che andrebbero discussi e approvati per cambiare una situazione economica assai grave e ovviare alla mancanza di politiche del lavoro e industriali, non possiamo non augurarci che il Governo e la maggioranza, in un sussulto di attenzione sui problemi concreti che riguardano i cittadini italiani, trovino il tempo e la voglia di affrontare questi temi. come ho detto, ha da tempo depositato varie proposte, e su cui naturalmente è pronto al confronto.

un orizzonte più sereno. Ma vi sono state anche alcune osservazioni, come sempre molto puntuali, da parte della collega Ghedini e del collega Nerozzi che credo meritino una puntualizzazione. Questo non è affatto un intervento minore, come lo si è voluto dipingere, quindi prefigurando la necessità di interventi strutturati e illuministicamente compiuti da parte della maggioranza. Questo è invece un provvedimento dietro il quale pulsa in maniera nitida la complessità del disegno di riforma legislativa di questa maggioranza. In primo luogo, si inserisce coerentemente dentro la traiettoria della sussidiarietà, che valorizza massimamente il ruolo, il contributo e l'apporto delle parti sociali e delle categorie professionali. È esattamente lungo questa traiettoria (che vuole dire meno legge e più contratto, più contratto aziendale e meno contratto nazionale) che questo provvedimento si inserisce, in qualche modo rievocando quella *big* *society*, quel meno Stato e più società, che si traduce, si invera e si materializza nella prevalenza data alla capacità autorganizzativa della categoria attraverso la previdenza. Addirittura si collega la flessibilità previdenziale alla qualità e all'intensità remunerativa della *performance* professionale. Tra l'altro, le parti sociali determineranno liberamente il posizionamento quantitativo del loro contributo, in relazione alla loro puntuale, specifica, concreta e prospettica condizione finanziaria e patrimoniale: questo vuol dire autonomia e valorizzazione dell'autonomia delle parti sociali! Abbiamo accolto molto volentieri la raccomandazione proposta dall'amico e collega Vaccari. Ma attenzione: guai se si tornasse a una sorta di forzosa omologazione: tutti al 4, al 5 o al 3. No, ciascuna cassa in relazione alla sua

di una riforma complessiva dell'economia e della società, che non a caso la maggioranza sottolinea appartenere alla tradizione culturale dell'economia sociale di mercato o, per dirla con un termine più schietto, ad un modello neocorporativo: ovviamente, il modello neocorporativo della scuola di Friburgo, non quello di

perché il centro, il *focus* non è il cittadino consumatore, bensì il cittadino produttore di beni e servizi, organizzato nella dimensione della sua associazione di rappresentanza professionale.

al centro di questa riforma, che tutto è salvo che una riforma minore: come riforma non minore ma decisiva. Noi la votiamo in modo compiuto e convinto.

Da un'indagine conoscitiva della Commissione bicamerale sugli enti gestori, risulta che l'ENASARCO, la cassa che dovrebbe garantire la pensione agli agenti di commercio, ha la maggiore esposizione indiretta in titoli Lehman per un controvalore di 780 milioni di euro; l'ENPAIA, la cassa degli agricoltori, 45 milioni;

la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina,

nella giornata di domani verrà posto all'ordine del giorno il seguito della discussione dei disegni di legge sulle squadre investigative comuni sovranazionali, per i quali la Commissione bilancio ha rettificato il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso il 2 marzo scorso. Il calendario della settimana sarà integrato con un'informativa del Ministro dell'interno sulla questione dei flussi migratori provenienti dal Nord Africa, auspicabilmente giovedì mattina. Giovedì pomeriggio si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata con ripresa diretta televisiva. Il ministro dello sviluppo economico Romani risponderà a quesiti riguardanti la politica energetica nazionale. Nel corso della prossima settimana, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, il calendario prevede l'esame del disegno di legge recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, il seguito della mozione Micheloni sulla razionalizzazione della rete diplomatico-consolare italiana, nonché la mozione Finocchiaro sugli stabilimenti balneari. Nella seduta antimeridiana di mercoledì 13 aprile, alle ore 9,30, il Ministro per i beni e le attività culturali renderà un'informativa sulle linee programmatiche del suo Dicastero. La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre convenuto che il decreto-legge recante disposizioni sulla cultura e altre disposizioni urgenti sarà posto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di lunedì 18 aprile. In tal modo, l'esame del decreto potrà concludersi prima delle festività comprese tra la Pasqua e la Festa del Lavoro, potendosi fin d'ora prevedere che in quella settimana l'Assemblea non terrà seduta.

che domani, 6 aprile, nella seconda ricorrenza del terremoto dell'Aquila, la seduta pomeridiana iniziasse con una commemorazione dei 309 morti

Presidente, considerando quanto il mio Gruppo ha rappresentato nella Conferenza dei Capigruppo, lo *speech* che lei ha letto poc'anzi funziona, tranne in un avverbio che sa di acqua fresca. «auspicabilmente» il ministro Maroni verrebbe nella giornata di giovedì. L'Italia dei Valori vota il calendario se viene espunta l'espressione «auspicabilmente».

egli già dovuto rinviare quella preannunziata per stamattina alla Camera, proprio perché impegnato in questa delicata e complessa missione tunisina. Sicuramente, però - non auspicabilmente o verosimilmente - la missione completerà il suo *iter* al massimo nella giornata di domani, mercoledì.

sia messo nelle condizioni di poter svolgere un minimo di attività di di collaborazione, di confronto e di sostegno alle ragioni del Governo, qualora le ritenesse fondate.

In sostanza, non voteremo questo calendario se non avremo la certezza che giovedì mattina il Ministro parteciperà ai lavori del Senato informando il Parlamento di ciò che ha fatto Tunisi e di quali

se il Ministro dovesse prolungare la sua visita in Tunisia fino a giovedì, potremmo sentire il ministro Fitto, che almeno sulla parte relativa

gli insegnanti e gli allievi dell'Istituto comprensivo «Luigi Pirandello» di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. *(Applausi)*.

per manifestare la nostra solidarietà alle agenti di polizia penitenziaria che hanno indetto uno sciopero della fame e del sonno all'interno della struttura, senza mai rientrare nelle loro abitazioni, per denunciare le gravi carenze di organico. «Lo sciopero» - dicono in una lettera inviata al direttore del carcere ed alla stampa - «si protrarrà fino a quando non sarà assicurato un incremento adeguato e doveroso del personale femminile». Le agenti sottolineano che la situazione lavorativa è diventata davvero insostenibile per carichi e turni di copertura, divenuti sempre più pesanti sia della carenza di personale, sia del sovraffollamento, e tutto ciò con gravi ricadute anche sulla loro vita familiare ed affettiva. «Siamo allo stremo delle nostre forze.» - denunciano le agenti - «Accusiamo demotivazione lavorativa, anche perché, guardando al futuro, vediamo solo incertezze, se non addirittura indifferenza e promesse vane da parte degli organi competenti». E concludono il comunicato dicendo: «Stanche sì, rassegnate mai».

nessuna risposta positiva da parte del Governo. Vorrei invitare dunque il ministro Alfano a smetterla di fare dichiarazioni di intenti e a passare davvero dalle parole ai fatti. Speriamo che lei, signora Presidente, possa riferire al Ministro questa nostra richiesta.

e della piccola e media impresa) ha lanciato un allarme preoccupante per le aziende piemontesi, che continuano ad investire, nonostante tutto, nelle energie rinnovabili. Il Presidente della CNA ha lanciato questo allarme molto preoccupato perché a causa dei pesantissimi tagli fatti dal Governo in materia di energie rinnovabili

e quindi mette concretamente a rischio tantissime piccole imprese che stanno lavorando in questo settore e che occupano, solo nella Regione Piemonte, circa 15.000 addetti. Secondo la CNA, come viene riportato dagli articoli se il provvedimento governativo sarà confermato - e purtroppo, ad oggi, non abbiamo segnali di diversa natura - in Piemonte sono a rischio migliaia di posti di lavoro. Credo, signora Presidente, che questo appello, che riguarda la mia regione, tocchi un tema che riguarda tutta l'Italia,

i Carabinieri, l'ambulanza e i Vigili del fuoco sono stati fatti andare via. Pertanto, vorremmo sapere dal Ministro dell'interno e dal Ministro delle attività produttive (al quale

a nome dell'intero Senato della Repubblica, degli auguri di pronta guarigione a questo nostro ufficiale così vilmente colpito da un attentato.

risposta ad alcune interrogazioni riguardanti le casse di previdenza. È stato appena approvato, con il mio voto contrario, l'aumento dal 2 al 5 per cento dei

vendita a Roma, in particolare da ENASARCO e dalla Cassa dei ragionieri, che metteranno in mezzo alla strada le famiglie che non si potranno permettere di acquistare quelle case che hanno abitato per tanto tempo. tempo. Ricordo, signora Presidente, che qualche anno fa, quando ci fu lo scandalo dei cosiddetti "furbetti del quartierino", l'ENASARCO, allora del presidente Sergio Billè, mise in vendita il patrimonio immobiliare secondo una valutazione di 3,5 miliardi di euro; questo quando doveva essere venduto agli immobiliaristi amici.

delle stesse casse e le future pensioni, con perdite rilevanti e che del resto anche i collegi sindacali delle casse stesse non sembra abbiano assolto all'obbligo di una verifica preventiva sulla rischiosità dell'investimento e sui proponenti, probabilmente ubicati presso il paradiso fiscale delle isole Cayman. scusa se ritorno sempre su questi argomenti, ma il compito di un senatore penso sia anche quello di difendere gli interessi e i diritti

di questi amministratori, che non hanno fatto nulla per evitare di mettere a repentaglio le future pensioni. La ringrazio molto per la sua sensibilità. per portare all'attenzione della Presidenza del Senato una situazione estremamente delicata. Questa mattina mi sono recata al centro di accoglienza di Santa Maria Capua Vetere, dove nella giornata di ieri sono stati trasferiti 500 migranti sbarcati al porto di Napoli, accompagnata da un mediatore culturale indicato dal prefetto di Napoli, che già ieri aveva accompagnato quei giovani.

Ho potuto avere informazioni dal campo da parte di suor Rita Giaretta, che conosco bene per il suo impegno, la quale ha accesso al campo. Mi sono chiesta se, vestendomi da suora, potevo entrare anch'io come parlamentare.

Questo è grave, è un precedente gravissimo. Si tratta peraltro di un carcere militare e non è affatto chiaro per quale motivo una struttura di identificazione debba essere collocata dietro porte blindate e perché questo sia stato possibile. Il ministro Maroni risponderà a tal riguardo, ma chiedo comunque alla Presidenza di farsi carico di questa istanza, perché analogo trattamento hanno ricevuto altri parlamentari a Manduria e negli altri centri recentemente